Signora Presidente, il motivo che ha dato origine a questa interrogazione è una notizia di stampa.

devono essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria». La norma del 2009 sancisce, 2009 sancisce, altresì, che: «Saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi». Evidentemente, anche scambiare oggetti e cuocere cibi è ritenuto motivo di preoccupazione. prevede che «l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna» abbia l'obiettivo di «prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate», alleate», si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo ritenga legittimi gli incontri di esponenti di primissimo rilievo della criminalità organizzata, all'interno di strutture penitenziarie preposte alla permanenza di soggetti sottoposti sottoposti al regime detentivo speciale; se non ritenga che situazioni analoghe a quelle di cui in premessa - ove effettivamente accertate possano rischiare di compromettere le azioni di contrasto alla criminalità organizzata poste in essere sia dalla magistratura che dallo stesso Ministro della giustizia, anche alla luce del potere conferitogli dal comma 1 dell'articolo 41-*bis* citato, consistente nella facoltà di sospendere l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati, nel quadro di quanto disposto dalle vigenti norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale. per non occupare troppo tempo, resta pendente l'osservazione critica che, mentre il Governo e la maggioranza sostengono continuamente di esercitare un'azione significativa

personaggi di sicuro spessore criminale, che potrebbero approfittare di queste condizioni di lassismo per portare a compimento altri disegni criminosi.

Faccio presente, infatti, che l'ordinamento penitenziario, come da ultimo modificato dalla legge n. 94 del 2009, prevede, tra l'altro, che ai detenuti sottoposti al regime detentivo speciale di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario venga assicurata la fruizione di momenti di socialità, all'interno di gruppi composti da non più di quattro elementi. Nell'ambito di tale normativa vanno inquadrate, quindi, le disposizioni impartite dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, in esecuzione delle determinazioni assunte dalla competente autorità giudiziaria. In proposito, tengo a precisare che l'assegnazione del detenuto Schiavone Francesco presso la casa di reclusione di Milano Opera fu disposta previa indicazione della direzione distrettuale antimafia di Napoli, la quale, alla luce degli sviluppi investigativi, aveva segnalato l'esigenza di intervenire, procedendo ad una diversa dislocazione degli esponenti di vertice del *clan* dei casalesi, per impedire che costoro continuassero ad esercitare dai carcere il loro ruolo direttivo nella gestione delle attività criminali. Peraltro, sia il trasferimento del detenuto Schiavone, sia la composizione del gruppo di socialità insieme al detenuto Graviano Giuseppe furono individuati nel corso di una riunione svoltasi presso la procura nazionale antimafia tra la predetta autorità giudiziaria e la direzione distrettuale antimafia di Palermo. Tutte le decisioni furono assunte preventivamente per assicurare la concertazione di ogni singolo aspetto dell'operazione e furono in seguito comunicate al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per assicurare la movimentazione prevista. Nella sede di nuova assegnazione, il detenuto Schiavone Francesco fu sottoposto dal 9 agosto 2008 al 6 maggio 2009 - su richiesta della direzione distrettuale antimafia di Napoli ed in costanza del regime speciale del 41-*bis* - anche alla sorveglianza particolare cui all'articolo 14-*bis* dell'ordinamento penitenziario, con il conseguente divieto di qualsiasi contatto con gli altri ristretti. Inoltre, dal 14 febbraio 2009 al 14 agosto 2009 al predetto detenuto fu fatta espiare anche la pena accessoria dell'isolamento diurno. Ciò posto, gli unici periodi in cui i detenuti Graviano e Schiavone fruirono congiuntamente della prevista socialità vanno dal 22 giugno 2008 al 9 agosto 2008, dal 15 agosto 2009 al 25 settembre 2009 e, infine, dal 22 dicembre 2009 al 2 gennaio 2010. Ad ogni buon conto, vorrei segnalare che la competente direzione generale dell'amministrazione penitenziaria ha ritenuto, all'indomani dell'annullamento dell'isolamento diurno per il detenuto Graviano, di procedere ad una diversa allocazione dei reclusi in regime di 41-*bis*, presenti nella casa di reclusione di Milano Opera. In data 3 gennaio 2010 veniva disposta, infatti, una diversa distribuzione dei suddetti reclusi all'interno dei posti disponibili nelle aree riservate dell'istituto. La scelta veniva prontamente comunicata alla procura nazionale antimafia ed alle direzioni distrettuali antimafia di Caltanissetta, Napoli e Palermo, ai fini della richiesta ratifica. Da quella data, dunque, i detenuti Francesco Schiavone e Giuseppe Graviano sono stati ubicati in spazi diversi e senza possibilità di incontro. Attualmente, il Graviano trascorre i momenti di socialità normativamente previsti con un altro detenuto, parimenti sottoposto al regime speciale; lo Schiavone, invece, è allocato da solo poiché dal 10 febbraio 2010 sta espiando un ulteriore periodo di isolamento diurno, della durata di due anni.

in parte. Se ho capito bene, il periodo di rapporto reciproco tra questi due personaggi è stato assai più lungo e ripetuto di quanto io supponessi in base alle informazioni di stampa.

contatti impropri tra soggetti che dovrebbero essere tenuti accuratamente separati, mentre, invece, a quanto risulta da ciò che riferisce il Sottosegretario, questi contatti sono stati ripetuti a cadenze cicliche. Restano pertanto motivi di forte preoccupazione.

tenuto conto che le questioni contenute nelle interrogazioni parlamentari in esame, alle quali si risponde congiuntamente, rientrano nella competenza locale, espongo gli elementi informativi di competenza della Regione Lazio, acquisiti per il tramite dell'ufficio territoriale del Governo di Roma L'azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma ha precisato di aver adottato gli atti deliberativi citati nelle interrogazioni parlamentari, riguardanti il conferimento di incarichi dirigenziali e l'indizione di bandi di selezione interna riservati al personale dipendente dell'azienda, per l'affidamento temporaneo di incarichi di responsabile facente funzioni di unità operative

prevista dall'atto aziendale approvato in data 3 aprile 2007 e successivamente modificato con deliberazione del 12 ottobre 2007, in linea con gli indirizzi regionali e conformemente alla normativa vigente in materia, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 6 al bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 35, del 20 dicembre 2007. A tale riguardo, si osserva in via preliminare che gli incarichi assegnati dal direttore generale dell'azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata non sembrano configurarsi come nuove assunzioni ma, appunto, come incarichi assegnati a personale già in servizio. Gli atti in questione non sono stati sottoposti dalla Regione Lazio alla validazione dei Ministeri competenti, ma si precisa che è prevista entro il 31 ottobre la revisione degli atti aziendali, finalizzata alla riduzione del 10 per cento delle unità operative complesse, semplici e dipartimentali del personale della dirigenza, nonché delle posizioni organizzative e di coordinamento per il personale del comparto. Per quanto riguarda il conferimento di incarichi disposto dall'ASL RM/D, il commissario straordinario dell'azienda, a seguito di specifica richiesta rivolta dal dipartimento programmazione economica e sociale della Regione Lazio, ha precisato che «l'avviso di selezione interna, ai sensi dell'articolo 3-*sexies*, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 (...) per il conferimento di n. 4 incarichi, di durata quinquennale,

Tale avviso è stato pubblicato dalla Regione Lazio sul bollettino ufficiale della Regione n. 12 del 27 marzo 2010, ma non è mai stato espletato. Infatti, in osservanza ad apposite indicazioni regionali successivamente pervenute con la nota del subcommissario per l'attuazione del piano di rientro,

di direttore di struttura complessa. Dette assunzioni sono state autorizzate in deroga al blocco del *turnover* per l'anno 2009. Pertanto, il decreto di cui sopra ha ottenuto, conseguentemente, la validazione dai Ministeri competenti. Gli incarichi assegnati in data 29 marzo 2010, citati in una delle interrogazioni a cui si risponde, sembrerebbero dunque riconducibili alle autorizzazioni di cui al richiamato decreto n. 91 del 2009. Resta inteso che i Ministeri competenti proseguiranno nell'esercizio delle proprie competenze per verificare il rigoroso rispetto dei piani di rientro.

Non mi scandalizzo di questo, ma del fatto che un direttore generale in carica,

ben 40 incarichi professionali. Questo è lo scandalo. Una settimana prima di dover lasciare l'incarico per fine mandato, si provvede a riempire tutti i posti vuoti inventandoli ulteriormente. Mi permetterò, gentile Sottosegretario, di inviare questa interrogazione alla Corte dei conti per tutti gli atti che la Corte dei conti riterrà utili nel rispetto delle prerogative anche di coloro i quali volevano partecipare e non hanno potuto farlo e penso a tutti coloro che, essendo stati sotto ai 40 nominati, speravano di essere nominati.

allora commissario *ad acta*, che invitava i direttori generali a non fare nomine ulteriori: credo sia rimasta carta straccia. La ringrazio quindi per la cortesia della sua risposta, gentile Sottosegretario,

Signora Presidente, ringrazio il senatore Astore che permette, con questa interrogazione, di chiarire un caso che ha suscitato qualche perplessità quando è uscito sulla stampa nazionale. Il trapianto comporta profonde implicazioni psicologiche, esistenziali, affettive, relazionali e sociali sia per il candidato al trapianto che per il donatore vivente e la sua famiglia. Lo studio e la valutazione degli aspetti psichici sono di fondamentale importanza per evitare o, quantomeno, scongiurare che aspetti non adeguatamente considerati, possano con il trapianto determinare un disagio psichico e sofferenza psicologica per il paziente stesso. Sin dal 2005 le problematiche attinenti al trapianto e al relativo impatto sulle condizioni psicologiche e psichiatriche del paziente sono state oggetto di attenzione per il Ministero della salute. In questo contesto vanno viste sia le linee guida del Centro nazionale trapianti (CNT), finalizzate a definire le modalità e gli *standard* omogenei per prevenire o arginare eventuali complicanze psichiche *post-*trapianto, trasmesse agli assessori e alla rete trapiantologica nel giugno del 2005, sia tutta la formazione di un gruppo di esperti nelle discipline di psichiatria e psicologia dei trapianti, che attualmente si è costituito in società scientifica. La valutazione psicologico-psichiatrica è di particolare importanza per l'inserimento in lista di attesa per il trapianto di organi. L'inserimento, infatti, deve avvenire anche in considerazione di alcuni aspetti psicologici, di carattere generale, del paziente e del contesto relazionale all'interno del quale lo stesso vive. Tali criteri, lungi dall'essere selettivi, devono considerarsi parametri di valutazione da adottare in ogni singolo caso volti a garantire al meglio la salute del paziente. Nel merito della questione, si osserva che nel 2009 la Regione Veneto ha elaborato una linea di indirizzo che integra i criteri da utilizzare per la valutazione dei pazienti pre-trapianto. Nell'allegato A alla delibera di giunta regionale n. 851 del 2009 vengono citate le indicazioni e le posizioni, in materia, di diversi autori, ma va da subito chiarito che l'impianto e le principali indicazioni contenute nella citata delibera sono in linea con i principi e le valutazioni sopra esposti. In sostanza, si tratta di un allegato che cita le posizioni di diversi autori fornendo informazioni sul dibattito in questione. Va anche detto che, fino ad oggi, nella Regione Veneto sono stati trapiantati 28 bambini con ritardo mentale. In nessun caso sono state effettuate discriminazioni sulla base di indicazioni generali. A seguito di una interpretazione non in linea con i contenuti della delibera, riferita ad una pubblicazione scientifica citata, la Regione Veneto ha inteso adottare una circolare esplicativa dei contenuti della medesima delibera, proprio per fugare ogni dubbio e superare le difficoltà interpretative che si erano determinate. In particolare, tale circolare chiarisce che il «documento ha il significato di indicare ed evidenziare le condizioni nelle quali, per eseguire con successo il trapianto, è necessario mettere in atto interventi di tipo diagnostico e terapeutico, nonché una rete di sostegno, finalizzati a garantire il massimo delle possibilità di cura, anche in presenza di rischi aumentati». Il Ministero della salute, unitamente al CNT, condivide i contenuti della circolare esplicativa della Regione Veneto. Si segnala, da ultimo che la questione sarà posta, in accordo con quanto proposto dall'assessore regionale, anche alla Conferenza degli assessori, al fine di condividere gli indirizzi per unificare, a livello nazionale, i criteri di inserimento di persone affette da disabilità nelle liste d'attesa e l'attenzione verso eventuali problematiche *post*-trapianto. Tali attività seguiranno le indicazioni fino ad ora fornite alle Regioni dal CNT, anche in collaborazione con gli esperti che, come sopra riferito, dal 2005 si interessano di tali materie.

Sono felice che la Regione Veneto sia tornata indietro, ma alcuni tentativi di escludere il disabile dal trapianto credo ci siano stati. Del resto, la stampa nazionale in quei giorni - lei lo ha ricordato - ha illustrato ampiamente. Con la circolare esplicativa pare che si sia tornati indietro e si sia riportata la materia in un'ottica di ordine nazionale. Approfitto di questa occasione, cara Sottosegretaria, per sottolineare che questo Paese, l'Italia, credo sia uno dei Paesi più avanti nella cultura del trapianto (in base alle statistiche e così via), che io credo che la questione centrale, signor Sottosegretario (approfitto di questa occasione per i pochi minuti che ho per parlare chiaro, perché faremo le barricate su alcune questioni) come, nel rapporto Stato-Regioni-enti locali, cominciano ad elevarsi steccati tra le sanità regionali. Sono fautore del federalismo,

mi affido a questo Governo, l'ho ricordato anche al Presidente del Consiglio durante il dibattito sulla fiducia - credo debba rimanere un compito essenziale, quello di garantire i diritti ai di non limitarli soprattutto nel campo della salute. E che dire, per esempio, delle liste di attesa enormi in alcune Regioni, mentre in altre Regioni c'è la proibizione di andare in certi ospedali perché è terminato il *budget*? Queste sono cose che avvengono sotto gli occhi di tutti, tutti i giorni. Se qualcuno oggi si rivolge al San Raffaele - dico un nome per fare un esempio - o al Gemelli di Roma, spesso e volentieri si sente rispondere che è terminato il *budget*. Io credo che lo Stato debba stare attento a garantire un diritto uguale per tutti dalle Alpi alla Sicilia. Questo è essenziale per il federalismo. L'essenza stessa del federalismo è proprio l'uguaglianza nell'erogazione di alcuni servizi. È vero che la sanità deve essere di gestione regionale: benissimo, nella maniera più assoluta, ma i livelli essenziali di assistenza, vivaddio, sono e devono rimanere di esclusiva competenza dello Stato. Io credo che questo momento delicato

fermo restando l'*iter* dei decreti delegati sul federalismo, che non deve essere assolutamente fermato, avviassero un'altra riflessione globale e complessiva su quella che deve essere la più grande riforma dello Stato repubblicano. Va benissimo la

la sempre maggiore esigenza di medici rappresenta una problematica che è già da anni all'attenzione del Governo. Per l'anno accademico 2010-2011, in considerazione della prioritaria necessità di garantire agli studenti standard formativi di qualità, non è stato possibile, nell'ambito della programmazione del corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in particolare per quanto riguarda la determinazione dei posti, prevederne un numero maggiore di quello risultante dall'analisi della capacità strutturale delle singole università. In tal senso, quindi, si è provveduto a confermare l'offerta potenziale formativa deliberata da ciascun ateneo. In merito alla possibilità di individuare meccanismi di accesso sostitutivi di quello attuale, con particolare riferimento alla graduatoria nazionale proposta dalla senatrice Garavaglia nel proprio disegno di legge, Atto Senato n. 1943, «con il quale si delega il Governo a predisporre apposito strumento per amministrare lo stesso *test* in tutte le Università, lo stesso giorno e quindi poter stilare una graduatoria nazionale», si ricorda che, già negli anni accademici 2005-2006 e 2006-2007, tale graduatoria era stata introdotta, a livello sperimentale, per il solo corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria. Tale scelta operativa era stata dettata dal numero dei partecipanti alla selezione, più esiguo rispetto a quello relativo al corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia. L'esperienza maturata in quegli anni può dirsi positiva per quanto riguarda la valorizzazione del merito in riferimento alla generalità dei candidati sul territorio nazionale, come evidenziato dalla senatrice Garavaglia in riferimento ai limiti del sistema attuale. L'esperienza in questione non può tuttavia essere considerata altrettanto positivamente per ciò che riguarda l'interesse manifestato dagli studenti ai fini della successiva iscrizione: ognuno dei partecipanti in posizione utile per l'immatricolazione avrebbe infatti dovuto confermare in via informatizzata il proprio interesse e procedere in tempi definiti alla relativa iscrizione. Purtroppo, in diversi casi l'iscrizione non è stata completata, o si sono verificate rinunce o passaggi ad altri corsi. Ciò ha determinato la necessità di rideterminare le posizioni in graduatoria, il tutto a detrimento della certezza delle successive immatricolazioni e dei tempi relativi alla conclusione delle operazioni che avrebbero consentito il regolare avvio dell'anno accademico. La complessità della procedura, ed in particolare la poca affidabilità da parte degli studenti in relazione alla scelta della sede, hanno evidenziato i limiti della graduatoria nazionale in questione ed hanno indotto l'amministrazione a non rinnovare la sperimentazione, tanto meno ad estenderla ad altre facoltà. Le criticità riscontrate, in particolare, sarebbero state certamente ancor più evidenti ed avrebbero influenzato pesantemente il buon andamento della procedura se applicate al corso di medicina e chirurgia, caratterizzato da una partecipazione senza dubbio più numerosa. Le proposte della senatrice Garavaglia potranno, comunque, essere valutate in sede di definizione delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi universitari a numero programmato o chiuso per l'anno accademico 2011-2012, essendo oramai conclusi i lavori relativi al prossimo anno accademico 2010-2011.

Sottosegretario emerge che non può essere contenta nemmeno l'amministrazione di come avvengono questi test.

immigrazione di medici da altre parti d'Europa o del mondo; esistono una cultura terapeutica, una capacità di rapportarsi ai nostri cittadini, una storia della medicina italiana, un suo umanesimo e un'antropologia medica che esigono che si pensi, e per tempo,

per incarichi e appalti importanti, figurarsi se non può attivarsi anche per stilare la graduatoria di tutti i giovani che partecipano al test. Una graduatoria nazionale non è molto diversa dalle graduatorie con cui assumiamo gli insegnanti: per eliminazione, quando un giovane si ritira, subentra il successivo, sapendo tutti

Il ministro Gelmini, ad un certo punto, accolse un emendamento, ma il Gruppo della Lega lo rifiutò, temendo che avrebbe danneggiato i ragazzi del Nord. Incredibilmente, sarebbe stato utile ai ragazzi del Nord, come risulta dai dati del test*,* la maggior parte di coloro che hanno raggiunto risultati positivi sono del Nord. Se un'università del Nord ha

il quarantesimo trova la possibilità di fare il suo corso, mentre il trentunesimo del Nord no. Bisogna quindi guardare a questi eventi con la larghezza di idee e la generosità che esige il Paese. Abbiamo bisogno di medici e di medici preparati.

Ci troviamo, credo, di fronte ad un'occasioni importante: si sta discutendo la riforma universitaria, che ha una sua strada, ma in quella riforma la logica del merito, della valutazione del merito e del recupero di tutte le migliori qualità ed intelligenze del Paese, dovrebbe essere uno dei fondamenti. Credo si comincino ad onorare quei principi, anche attraverso la prova selezione che avvia i giovani alla facoltà di medicina e chirurgia. Voglio ricordare, da ultimo, signor Sottosegretario e colleghi,

Nell'interrogazione si fa presente che la Cofiloc Spa, società con sede in provincia di Treviso che svolge l'attività di noleggio di macchine ed attrezzature per lavori edili, ha ricevuto dal competente ufficio dell'Agenzia delle entrate un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2004 (impugnato presso la Commissione tributaria provinciale) ed è stata oggetto di verifica fiscale per i periodi d'imposta 2005, 2006 e 2007. Più in particolare, l'ufficio contesta alla Cofiloc Spa l'errata applicazione dei coefficienti di ammortamento previsti dal decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 poiché la società, non essendo un'impresa edile bensì un'impresa di noleggio di macchine ed attrezzature edili, avrebbe dovuto applicare il coefficiente del 7,5 per cento previsto per il gruppo di «attività non precedentemente specificate» anziché quello del 15 per cento previsto per le «imprese di costruzioni edilizie». Di conseguenza, il recupero a tassazione ha riguardato i maggiori ammortamenti calcolati dalla società e i canoni di *leasing* relativi a gru e piattaforme aeree. Nell'interrogazione si sostiene che tale interpretazione è illegittima in quanto, in primo luogo, si porrebbe in contrasto con la *ratio* dell'articolo 102, comma 2, del TUIR e del decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 i quali prevedono che i coefficienti di ammortamento dei beni materiali strumentali «sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi». Nel caso di specie - secondo l'interrogante - non vi è dubbio che il settore produttivo al quale ricondurre il deperimento ed il consumo delle gru e delle piattaforme sia quello delle industrie edilizie e non quello delle altre attività anche perché tutti i beni strumentali oggetto dell'attività della Cofiloc Spa sono impiegati ed impiegabili soltanto nel settore dell'edilizia e tutti i clienti della società sono imprese edili. A sostegno della propria tesi l'interrogante richiama i principi espressi dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 13506 dell'11 giugno 2009 (la categoria a cui appartiene un bene ai fini dell'ammortamento deve essere individuata "utilizzando non un criterio meramente descrittivo(...) ma un criterio sostanziale") nella sentenza n. 5241 del 12 maggio 1995 ("il ricorso non è fondato, perché sorretto da argomenti di pura logica formale e ignaro, quindi, delle ragioni di ordine sostanziale che presiedono alla diversificazione dei coefficienti di ammortamento dei beni ammortizzabili, sicuramente incentrata sul variabile tasso di usura dei medesimi, determinato, questo, dagli impieghi cui essi sono singolarmente destinati"). Nell'interrogazione vengono inoltre richiamati alcuni documenti di prassi con cui 1'amministrazione finanziaria si è espressa sul tema. In particolare, l'interrogante evidenzia il principio enunciato dalla nota n. 483/E del 23 maggio 1996, in cui si è affermato che «tenuto conto della disposizione contenuta nell'articolo 67, comma 2, del TUIR, la quale dispone che i coefficienti di ammortamento sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi, si ritiene che nel caso di locazione di un bene il coefficiente di ammortamento applicabile sia quello del settore produttivo dell'impresa utilizzatrice». Inoltre, nell'interrogazione si mettono in evidenza i contenuti della risoluzione n. In proposito, l'interrogante evidenzia che la «destinazione definitiva» delle gru e delle piattaforme aeree in questione e il loro «naturale impiego da parte del possessore» è inequivocabilmente nel settore dell'edilizia. L'interrogante, pertanto, chiede di sapere se il Ministro dell'economia e delle finanze intenda intervenire al fine di verificare se l'operato dei funzionari dell'Agenzia delle entrate di Treviso sia conforme con la prassi del Ministero e la giurisprudenza e se ritenga opportuno uniformare l'attività di controllo e verifica degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate

n. 56/E del 9 aprile 2004 e nella circolare n. 10/E del 13 marzo 2006. La risoluzione n. 56/E del 2004, relativa alla determinazione del coefficiente di ammortamento applicabile ad un immobile concesso in locazione da una costituenda società immobiliare, che è citata dall'interrogante a sostegno della tesi dell'infondatezza dei rilievi effettuati dai funzionari dell'ufficio di Treviso, legittima, ad avviso dell'Agenzia, la correttezza dell'operato dei controllori. In tale risoluzione, infatti, è stato affermato che ai fini dell'ammortamento dell'immobile da concedere in locazione la società immobiliare (soggetto locatore) è tenuta ad applicare l'aliquota fissata per gli immobili strumentali di proprietà delle società immobiliari, non rilevando la circostanza che la società utilizzatrice del bene operi in un diverso settore di attività. Nella risoluzione viene richiamata la sentenza della Corte di cassazione n. 5241 del 1995 e, più in particolare, le «ragioni di ordine sostanziale che presiedono alla diversificazione dei coefficienti di ammortamento dei beni ammortizzabili», che «sono da ricercare nel variabile tasso di usura dei beni medesimi». A tal proposito, la risoluzione aggiunge anche che l'usura «presuppone una destinazione definitiva del bene al suo naturale impiego da parte del possessore» e che essa «non può essere determinata tenendo conto di un utilizzo provvisorio e straordinario dello stesso». L'Agenzia è pervenuta alle conclusioni che emergono dalla citata risoluzione considerando che i coefficienti fissati dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988, per esigenze di razionalità e di sistematicità del procedimento di ammortamento fiscale, esprimono un valore medio slegato da una determinazione analitica dell'effettivo deperimento subito dai beni per effetto del loro utilizzo nell'attività produttiva. Basti pensare alle complessità che si determinerebbero qualora prevalesse la diversa tesi interpretativa che emerge dall'interrogazione nel caso di beni dati in locazione nello stesso anno o in anni diversi a soggetti che operano in settori per i quali sono previsti coefficienti diversificati. Risulta evidente che in questi casi non si potrebbe in nessun modo assicurare la sistematicità del processo di ammortamento che, invece, risponde ad esigenze di certezza volte ad evitare possibili arbitraggi da parte dei contribuenti. Tale orientamento è stato confermato anche nella circolare n. 10/E del 13 marzo 2006

richiede che si applichino i coefficienti del settore di attività riferibile a questi ultimi, prescindendo dall'effettivo utilizzo di tale bene o dalla sua eventuale locazione a terzi. Si pensi al caso dell'immobile condotto in *leasing* da una società immobiliare e dato da questa in locazione ordinaria ad un terzo che opera nel settore delle "industrie estrattive di minerali metalliferi e non metalliferi" La verifica della durata del contratto di locazione finanziaria andrà effettuata nella misura del 3 per cento, corrispondente al coefficiente di ammortamento previsto per gli edifici del settore "altre attività", a cui deve essere ricondotta l'attività della società immobiliare, e non in base al coefficiente del 5 per cento stabilito per i fabbricati destinati alle predette industrie». Nel caso prospettato dall'interrogante, il bene è evidentemente destinato in via definitiva all'attività di noleggio esercitata dalla Cofiloc (possessore) e non a quella edile della società cliente (detentore). Più in generale in caso di locazione/comodato a terzi di beni materiali strumentali, ai fini della corretta determinazione dei coefficienti di ammortamento applicabili rileva, quindi, l'attività esercitata dal locatore/comodante e non il settore di attività in cui il locatario/comodatario utilizza il bene. Tale interpretazione è anche coerente con i principi espressi nella sentenza della Corte di cassazione n. 13506 del 2009, citata nell'interrogazione, che riguarda il caso di una società che commercia apparecchiature elettromedicali che in parte vengono noleggiate a terzi (presumibilmente ad operatori del settore sanitario). In tale fattispecie la Cassazione, in relazione ai beni noleggiati, ha ritenuto applicabile il coefficiente del 25 per cento relativo ad una voce del «gruppo di attività non specificate» (in cui rientra l'attività di commercio del noleggiante), mentre - al contrario - ha escluso l'applicazione dell'aliquota del 12,5 per cento relativa alla voce «attrezzatura specifica», iscritta nel gruppo XXI Servizi sanitari (a cui presumibilmente appartiene l'utilizzatore dell'apparecchiatura elettromedicale). Se avesse voluto dare rilevanza all'attività esercitata dall'utilizzatore, la Cassazione non avrebbe confermato l'applicabilità dell'aliquota "residuale" del 25 Per tali ragioni, l'Agenzia delle entrate ritiene che il comportamento dei funzionari dell'ufficio di Treviso sia coerente con la prassi ufficiale più recente dell'Agenzia e con la giurisprudenza. suesposti principi deve tener conto di alcune situazioni di fatto nelle quali l'applicazione di un determinato coefficiente non rifletta l'effettivo deperimento del bene. È il caso - ad esempio - dei beni appartenenti a soggetti rientranti nel gruppo «attività non precedentemente specificate» quali - appunto - le imprese di noleggio, per i quali il coefficiente di ammortamento, che consente dì dare una rappresentazione più realistica del deterioramento, deve essere ricercato nel gruppo di attività dell'utilizzatore, in considerazione delle caratteristiche intrinseche del bene che - di fatto - comportano un utilizzo esclusivo in uno specifico settore di attività. Tale deroga ai principi generali può trovare applicazione solo a condizione che il bene venga impiegato per tutta la sua vita utile, esclusivamente nel medesimo settore di attività, anche da parte di più utilizzatori. In tal modo vengono comunque garantite, mediante l'applicazione di un coefficiente unico, la certezza e la sistematicità del processo di ammortamento, scongiurando anche il pericolo di possibili arbitraggi da parte dei contribuenti. Nel caso di specie, quindi, considerato che il bene strumentale viene dato in noleggio per la sua intera vita utile a soggetti operanti nel medesimo settore di attività, potrà trovare applicazione il coefficiente di ammortamento previsto con riferimento all' attività svolta dal locatario.

direzione secondo cui il coefficiente di ammortamento dell'impresa allocataria deve essere lo stesso dell'impresa destinataria.